Signor Presidente, signor Sottosegretario, il senso dell'interpellanza, presentata dal sottoscritto e da numerosi colleghi di maggioranza e opposizione, vuole sottolineare al Governo il caso della chiusura della redazione romana di Telepace, la cosiddetta TV del Papa.

posto, abbiamo avvertito l'esigenza e il sentimento di sottoporre al Governo l'opportunità di intervenire immediatamente su eventi che ormai si sono consumati, perché abbiamo presentato questa interpellanza nel momento in cui, a

che ha un valore essenziale e che ha portato alla ribalta eventi di carattere internazionale. Ebbene, questi giornalisti sono stati drasticamente e, a nostro parere senza una decisione motivata, licenziati.

sulle spese realmente sostenute nell'ultimo periodo da Telepace, ma soprattutto sulla vicenda, che non possiamo accettare, del licenziamento, a nostro avviso senza alcuna ragione, dei giornalisti Piero Schiavazzi, Angela Ambrogetti, Simona De Santis ed Elisabetta Mancini, nonostante il loro costante impegno e la loro bravura professionale avessero reso celebre in tutto il mondo la piccola emittente - italiana, non vaticana, vorrei sottolinearlo al rappresentante del Governo - con *scoop* a ripetizione, contribuendo così, in modo decisivo, a proiettare un'immagine della Chiesa, a Roma e altrove, estremamente aperta e positiva. Stranamente i responsabili di questa emittente sono rimasti sordi alle interrogazioni parlamentari e a tutti gli appelli lanciati - signor Presidente, anche lei ha sottoscritto la presente interpellanza in questi mesi da deputati, senatori, intellettuali, consiglieri regionali e comunali per bloccare il licenziamento. Io dico: peccato, si è persa un'occasione per trovare una soluzione intelligente, non l'arroganza che riscontriamo negli atteggiamenti

di avere imposto il timbro del cartellino ai giornalisti licenziati, in violazione del loro contratto nazionale di lavoro; di avere imposto un filtro alle telefonate in redazione, in violazione della legge istitutiva dell'ordine dei

che gli ispettori del Ministero del lavoro hanno rilevato e sanzionato, con 14.000 euro di multa, la violazione della legge che impone anche a Telepace l'obbligo di assumere un disabile;

che li ha sostanzialmente denigrati, facendo capire che non erano nel vero e rendendo noto che le ispezioni dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani si sono concluse con un addebito a Telepace pari a ben 70.000 euro per contributi evasi e a 20.000 euro di sanzioni.

testimonianza. Signor Sottosegretario, lei capisce quanto sia importante per noi conoscere che tipo di interventi il Governo voglia attuare per assicurare

Non voglio parlare di questioni giuridico-sindacali, voglio soltanto, con queste poche parole, rappresentare al Governo

le emittenti a carattere comunitario - tipologia cui appartiene l'Associazione Amici di Telepace - sono tenute all'osservanza di quanto previsto nella delibera n. 78/98 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi cui sono assoggettate le varie tipologie di emittenti. La delibera non impone per le emittenti del tipo in questione alcuna indicazione relativamente al numero e alle qualifiche dei lavoratori occupati. Tali elementi hanno invece rilievo per l'attribuzione del punteggio ai fini dell'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448 del 1998. In proposito, il decreto ministeriale n. 292 del 2004 indica il punteggio da attribuire ai diversi elementi, fra i quali è annoverato il personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, distinto per categorie e tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, *full time* o *part-time*). L'emittente Telepace (dell'Associazione Amici di Telepace) ha conseguito per l'anno 2005 una valutazione che ha tenuto conto della presenza, fra gli altri, di tre giornalisti professionisti e tre giornalisti pubblicisti occupati a tempo parziale, come risultante dal prospetto dei relativi contributi previdenziali versati, che hanno consentito all'emittente stessa di occupare un'elevata posizione nella graduatoria e di accedere al beneficio. Le risultanze del sopralluogo congiunto, effettuato dalla competente Direzione provinciale del lavoro di Roma e da funzionari di vigilanza dell'Istituto nazionale previdenza giornalisti (INPGI), hanno evidenziato irregolarità nel versamento dei contributi dovuti all'INPGI, derivanti, fra l'altro, dalla circostanza che alcuni giornalisti professionisti, pur risultando assunti *part-time*, svolgevano un orario di lavoro settimanale corrispondente a quello previsto per i rapporti di lavoro a tempo pieno. Tale inadempienza non ha però influito sulla determinazione ed attribuzione del punteggio finalizzato all'erogazione dei contributi previsti per le emittenti locali, in quanto la valutazione del personale dipendente da parte dei Corecom incaricati di accertare la sussistenza dei requisiti e predisporre le graduatorie regionali da trasmettere al Ministero delle comunicazioni - era stata effettuata sulla base della dichiarazione dei contributi previdenziali versati, riferiti a personale assunto *part-time*. Essendo il punteggio commisurato alle tipologie di impiego e al numero di dipendenti dichiarati, se l'emittente non avesse commesso l'irregolarità summenzionata, sulla quale - come illustrerò in seguito - pende ancora giudizio, e avesse adeguato la relativa dichiarazione, avrebbe ottenuto un punteggio ancora maggiore. La descritta situazione, quindi, pur sanzionabile sotto il profilo previdenziale, non dà titolo alla revoca dei contributi corrisposti all'emittente sulla base delle dichiarazioni effettuate. Per quanto concerne la programmazione, si fa presente che l'emittente Telepace di Roma ripete integralmente sul satellite (Eutelsat 13° est) le proprie trasmissioni via etere terrestre; ciò tuttavia non contrasta con le vigenti disposizioni, che consentono alle emittenti concessionarie o autorizzate di ripetere la propria programmazione su altra piattaforma di diffusione (satellite) senza la necessità di ottenere alcuna autorizzazione. Diverso è il caso di emittenti televisive che ripetono in contemporanea lo stesso programma (anche se satellitare), in quanto tale attività è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni che provvede, entro un mese dalla data del ricevimento della domanda, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005); in proposito, non risulta essere stata prodotta alcuna domanda da parte di alcuna emittente. L'accertamento di eventuali violazioni rientra nella competenza dell'AGCOM, che il Ministero delle comunicazioni solleciterà affinché intervenga per le verifiche del caso. Qualora esse appurassero la ripetizione del medesimo programma in contemporanea, effettuata in mancanza della domanda di relativa autorizzazione, ciò contribuirebbe ad avvalorare la percezione dell'organicità editoriale tra le varie emittenti, operanti in diversi bacini, che sono già individuate dal pubblico con la generica comune denominazione di Telepace. La questione riguardante le spese sostenute per l'affitto dei satelliti, come qualsiasi altra voce di costo sostenuta dalle emittenti per l'espletamento della propria attività, non può essere accertata, trattandosi di aspetti di natura privatistica ed afferendo all'attività di un'associazione non riconosciuta e quindi non tenuta a redigere un bilancio ufficiale. Il Ministero del lavoro e della previdenza, che abbiamo sentito in merito alle questioni segnalate dagli onorevoli interpellanti, dopo aver comunicato quanto già riferito in merito all'assunzione di giornalisti *part-time*, che, tuttavia, risultano applicati a tempo pieno, ha precisato che nel corso dell'accertamento effettuato dal competente servizio ispezione del lavoro, nella sede di Roma dell'Associazione Amici di Telepace, nel periodo 23 febbraio-4 maggio 2005, sono state raccolte le dichiarazioni spontanee del personale al momento applicato, composto da nove unità di tecnici e/o amministrativi e quattro unità di giornalisti, tutti risultati registrati sui libri obbligatori. Nell'occasione, il suddetto servizio ha rilevato e sanzionato la violazione della legge n. 68 del 1999 sul collocamento dei lavoratori disabili; l'Associazione, infatti, non aveva inviato al Centro per l'impiego di Roma il prospetto recante il numero di lavoratori occupati dal 2000 al 2005. I giornalisti hanno riferito di ritardi, anche notevoli, nel rilascio dei prospetti mensili di retribuzione che, tuttavia, da qualche mese venivano consegnati con regolarità; il personale tecnico, al contrario, ha dichiarato di aver sempre ricevuto regolarmente i predetti prospetti, comprendenti anche le eventuali ore di straordinario lavorate. Relativamente ai giornalisti professionisti utilizzati a tempo pieno, ma assunti *part-time* e per i quali sono stati versati i corrispondenti contributi previdenziali, sono stati richiesti i contributi effettivamente dovuti. In merito In merito alla vicenda è attualmente pendente, presso la sezione lavoro del tribunale di Roma, un giudizio di cognizione ordinaria sul merito delle contestazioni mosse, avendo la stessa Associazione Amici di Telepace proposto opposizione al decreto ingiuntivo che l'INPGI aveva chiesto e ottenuto dalla suddetta sezione lavoro del tribunale di Roma, relativamente all'importo dei contributi non regolarizzati a seguito dell'iniziale contestazione. Quanto all'emittente Telepace, della Fondazione artigiani della pace con sede a Verona, la locale Direzione provinciale del lavoro ha comunicato che la struttura giornalistica della stessa è composta da un capo redattore (nominato il 2 novembre 2004) e da cinque redattori (giornalisti), tutti assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato: i problemi si pongono soprattutto a Roma più che a Verona. Il servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Roma, nel comunicare di non aver ricevuto, durante la visita ispettiva, alcuna informazione da parte dei giornalisti della redazione romana in merito alle ritorsioni e agli abusi denunciati dall'Associazione Stampa Romana, ha fatto presente, relativamente alle esigenze economiche addotte quale motivazione per la chiusura della redazione giornalistica di Roma, che è stata fornita la situazione patrimoniale e il conto economico dell'Associazione Amici di Telepace solo ripeto solo - per il periodo 1° gennaio 2005-30 giugno 2006. Lo stesso servizio ispettivo ha inoltre evidenziato che, trattandosi di associazione non riconosciuta, per Amici di Telepace non è obbligatoria la redazione di un bilancio ufficiale. Risulta pertanto non procedibile una contestazione dei criteri di ripartizione degli importi introitati tramite donazioni e lasciti. Il Governo non può a tal proposito disporre di elementi di conoscenza aggiuntivi. Il Ministero della giustizia, da parte sua, nel confermare che, in merito ai fatti riferiti nell'atto ispettivo in esame, sono stati inoltrati alcuni esposti all'Ordine dei giornalisti del Lazio e che è stata avviata un'indagine da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha sottolineato che tali organi agiscono nell'ambito delle proprie autonome prerogative e attribuzioni, in merito alle quali il Governo non può interferire con specifiche richieste di informazioni, stante la stante la normativa vigente in materia. In tal senso, anche la procura della Repubblica di Roma, interessata al fine di ottenere informazioni, ha comunicato che gli elementi desumibili dall'interpellanza non consentono l'effettuazione di ricerche utili nel registro generale per individuare eventuali procedimenti penali iscritti. Pur nel dovuto rispetto dei limiti posti all'operato del Governo dalle vigenti normative, desidero informare gli onorevoli interpellanti e quest'Aula che, condividendo condividendo la preoccupazione per la situazione che ha colpito la redazione romana di Telepace e l'intenzione di favorire il miglior esito possibile a riguardo, sono state intraprese iniziative volte a promuovere una mediazione che possa assecondare una ricomposizione della controversia tra le parti. È stata ricevuta, a tal fine, una delegazione dell' Associazione Stampa Romana e della redazione di Telepace e sono stati allacciati contatti con la direzione dell'emittente in vista di un incontro che, nel rispetto dell'autonomia gestionale riconosciuta all'emittente, contribuisca a raccogliere ogni elemento utile che incoraggi un approccio costruttivo tra le parti nel comune impegno verso una soluzione che preveda la riconsiderazione dei provvedimenti di licenziamento.

e poi gli chiederò di aderire, nel suo stesso interesse, a partecipare ad una riunione (i cosiddetti «tavoli»), in cui ci sono le varie parti e in cui si cerca tutti insieme, con buona volontà, di trovare una soluzione al problema. Ho contattato anche il mio corrispondente del Vaticano e certamente il Vaticano è completamente estraneo

non è gradita, e quindi è interesse di tutti fare uno sforzo, trovarsi intorno ad un tavolo e trovare una soluzione condivisa. Io sono ottimista e mi auguro che si possa riuscire in un tempo ragionevole a risolvere, almeno in parte, questo problema.

mi rende fiducioso nell'azione del Governo e sua personale affinché la soluzione di questo problema sia una soluzione ovviamente illuminata, non muscolare,

Occorre innanzitutto ricordare che il decreto legislativo n. 79 del 1999 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di dare indirizzi operativi e strategici per il conseguimento dell'oggetto statutario della SOGIN S.p.a, mentre la competenza sui profili ispettivi delle attività operative della stessa SOGIN è attribuita all'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici). L'APAT, infatti, ha avviato una regolare istruttoria per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità relative al malfunzionamento verificatosi durante le prove di collaudo dell'impianto anti-incendio asservito ai locali 9 e 10 dell'impianto Plutonio ubicato nel centro di ricerca Casaccia dell'ENEA, ma gestito dalla SOGIN S.p.a. Il Ministero dell'ambiente ha comunicato, a riguardo, che nell'ambito dell'*iter* per il rilascio del certificato di prevenzione incendi per l'impianto Plutonio, i Vigili del fuoco hanno richiesto l'installazione di nuove serrande tagliafuoco sulle tre linee di mandata del sistema di ventilazione dell'impianto. Ad installazione ultimata, è iniziato il collaudo funzionale dei nuovi componenti. Il collaudo prevedeva una simulazione di incendio nei vari locali con la verifica della sequenza degli interventi dei dispositivi di azionamento ed interblocco. Il collaudo veniva svolto per i differenti locali sulla base delle procedure normalmente applicate dal personale dell'impianto negli interventi di manutenzione e nelle prove periodiche. Dette procedure prevedono che nelle fasi di prove sia esclusa la scarica dell'estinguente. In data 30 ottobre, il programma era pressoché terminato. Rimaneva da eseguire la prova del locale 9, il locale di deposito. Nel corso della prova, sebbene fosse stato escluso l'intervento automatico del sistema di estinzione, per un guasto nella scheda di controllo del sistema antincendio relativo al locale 9 questa esclusione di fatto non è avvenuta causando così la scarica simultanea nel locale di 36 bombole di estinguente. La sovrapressione generatasi ha divelto la porta tagliafuoco posta tra il locale 9 e il corridoio di comunicazione con il corpo principale dell'impianto e provocato la rottura di tre porte adibite ad uscita di emergenza verso l'esterno poste nel corridoio di collegamento dei laboratori. Immediatamente dopo l'evento sono stati presi provvedimenti per ripristinare il contenimento statico chiudendo la porta di sicurezza del locale 9 e sigillando le porte di emergenza danneggiate. Si è provveduto, inoltre, al distacco materiale delle bombole di estinguente del locale 9. Le misure di contaminazione radioattiva effettuate all'esterno impianto nelle immediate vicinanze delle porte di emergenza hanno fornito valori non distinguibili dal valore di fondo. Le misure di contaminazione radioattiva effettuate nelle aree interne dell'impianto coinvolte dall'evento (locale 9 e corridoio) e, successivamente, nei laboratori hanno fornito valori equiparabili ai valori rilevati nelle periodiche misure svolte in base al programma di sorveglianza fisica della radioprotezione dell'impianto. Secondo quanto comunicato dall'ENEA, dai primi accertamenti fatti dalle squadre radiometriche dei Vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine prontamente intervenute sul luogo, nonché da controlli ambientali eseguiti dall'ENEA stesso, non risultano contaminazioni né nell'impianto interessato dal malfunzionamento, né all'esterno di esso. In particolare, il personale presente o sopraggiunto nelle aree, anche potenzialmente interessate dall'evento, è stato sottoposto al controllo della contaminazione esterna e all'analisi del muco nasale. Inoltre, il personale presente nel corridoio interessato dall'evento o nelle vicinanze è stato sottoposto, come intervento immediato e in via cautelativa, alle metodologie di controllo e di verifica a bassa energia. Questo esame consente di accertare in modo pronto se vi sia stata una contaminazione interna di un certo rilievo. Tutti gli esami hanno dato esito negativo. Avendo potuto escludere contaminazioni interne acute, gli accertamenti sanitari per i lavoratori sono proseguiti secondo quanto previsto dal programma di radioprotezione in uso presso l'impianto. A seguito dell'evento, la SOGIN sta svolgendo, oltre ad una manutenzione straordinaria dei sistemi di rilevazione, estinzione incendio e del sistema di valutazione, anche un riesame delle logiche di interconnessione dei suddetti sistemi. Il risultato delle analisi in corso potrebbe comportare la revisione delle procedure di prova nonché interventi di miglioria sui sistemi in questione e sulle logiche di interblocco e di attuazione. L'APAT, comunque, sta svolgendo una serie di accertamenti indipendenti dai quali, oltre ad eventuali violazioni, potrebbero emergere ulteriori indicazioni circa l'opportunità di intervenire sulle attuali procedure o sulle vigenti prescrizioni. Verifiche più generali sono state avviate sulle modalità di gestione da parte della SOGIN delle attività di conduzione degli impianti, ad evitare il ripetersi di eventi che, come quello in questione, si sono manifestati nel corso degli ultimi tempi. che questi episodi denotano una problematica della quale l'APAT e la SOGIN vorranno farsi carico

statutario della SOGIN Spa, mentre la competenza sui profili ispettivi delle attività operative della stessa è attribuita all'APAT. Aggiungo che nelle situazioni in esame sono intervenuti poi provvedimenti e poteri speciali conferiti attraverso un'ordinanza che avrebbe dovuto garantire interventi efficaci a tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'ambiente. Gli episodi purtroppo dicono che le cose non sono andate esattamente come avrebbero dovuto. I quesiti posti dall'interrogazione trattano, prioritariamente, i seguenti aspetti relativi alle attività svolte presso l'area disattivazione SOGIN Spa, ubicata nel centro ricerca Casaccia dell'ENEA: la bonifica delle scatole a guanti ubicate nell'impianto Plutonio e la bonifica dell'area OPEC-1. Sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e, in particolare, dall'APAT, si evidenzia quanto segue. Riguardo al primo aspetto, si rileva che nel corso di analisi di *routine* per la valutazione di eventuali ingestioni-inalazioni di radioisotopi, effettuate tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2006, previste dal programma di sorveglianza di radioprotezione dei lavoratori dell'impianto Plutonio, si sono verificati sette casi anomali. Le analisi eseguite, secondo quanto previsto nei protocolli di sorveglianza della radioprotezione dei lavoratori applicati dalla SOGIN Spa, adottavano la tecnica radiotossicologica della spettrometria degli escreti. Le valutazioni di dose efficace dovuta alla contaminazione interna sono state effettuate sulla base dei dati risultanti dalle analisi secondo protocolli internazionali riconosciuti. Le dosi efficaci calcolate sono risultate inferiori e solo in un caso circa uguali ad un millesimo di Syvert. A seguito della comunicazione dei risultati delle analisi inviata dal laboratorio, il datore di lavoro ne ha data informazione ai lavoratori interessati e l'impianto è stato messo in stato di «impianto in carico», sospendendo, pertanto, le attività in corso ed avviando un'indagine per accertare le cause dell'evento. I risultati dell'indagine mostrano che la causa più probabile sia da attribuire ad una contaminazione residua riscontrata sull'esterno di una «scatola a guanti». Successivamente, è stata avviata una campagna straordinaria di misure per verificare l'esistenza di eventuale contaminazione. Tale campagna è stata estesa a tutte le aree operative dell'impianto Plutonio. I lavoratori risultati positivi alle analisi sono classificati, ai fini della radioprotezione, come lavoratori esposti di categoria A per i quali la legge stabilisce un limite di dose efficace annua di 20 millesimi di Syvert. I valori di dose efficace valutati per l'episodio in questione non pongono particolari obblighi di segnalazione da parte del datore di lavoro in quanto nettamente inferiori ai limiti di legge. L'impianto Plutonio è autorizzato all'esercizio da una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Tenuto conto della definitiva cessazione delle attività nucleari, la licenza di esercizio autorizza esclusivamente le attività di messa in sicurezza propedeutiche al suo completo smantellamento e la gestione dei rifiuti derivanti da dette attività. In questo ambito la bonifica delle scatole a guanti, operazione peraltro già ampiamente svolta in passato, rientra tra le normali attività previste dalla vigente licenza di esercizio. I rifiuti prodotti sono, come stabilito dalle procedure in atto, confezionati e inviati al complesso di trattamento e gestione dei rifiuti radioattivi del centro della Casaccia gestito dalla Nucleco Spa. II gruppo operativo dell'impianto Plutonio è formato sostanzialmente da personale ENEA già in organico presso il suddetto impianto e trasferito con comando dall'ENEA alla SOGIN all'atto del trasferimento alla suddetta società della titolarità della licenza di esercizio. Si fa presente, inoltre, che sei dei sette lavoratori risultati positivi alle analisi sono lavoratori ENEA in comando alla SOGIN ed uno è invece dipendente SOGIN. Per quanto riguarda l'evento in questione, l'APAT ha svolto, nell'ambito dei compiti attribuiti dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, un'azione di polizia giudiziaria volta ad accertare la sussistenza di eventuali aspetti penalmente rilevanti. Gli esiti di questa azione sono di competenza della magistratura. Per quanto riguarda, infine, la zona denominata Area Waste-B dell'impianto OPEC-1 si informa che, per ridurre il rischio di possibili diffusioni di radioattività all'esterno della cella di calcestruzzo interrata, nella quale è collocato il serbatoio metallico da 22 metri cubi circa, sono stati estratti e confezionati, come rifiuti radioattivi, i materiali rimovibili presenti nella cella stessa. Si tratta, in particolare, di uno strato di magrone e di sabbia, presenti nella camera superiore della cella nonché di acqua e di fango, presenti nella sezione inferiore a contatto con il serbatoio. Sono stati, infine, ripetuti i rilievi geognostici utilizzando le perforazioni effettuate nel 2002. Anche in questo caso i risultati, come nel 2002, hanno escluso la diffusione di radioattività all'esterno della cella di calcestruzzo. Tra l'altro, come è noto, il nuovo assetto di vertice della SOGIN, reso snello e più operativo dall'ultima legge finanziaria, si è appena insediato e si troverà ad affrontare tutte le questioni e i problemi connessi ai compiti ad essa assegnati nel 1999, nel 1999, relativi allo smaltimento e alla gestione delle scorie del nucleare innanzi tutto con la messa in sicurezza dei detriti e la riconversione delle vecchie centrali atomiche ora chiuse. Dalle due interrogazioni emerge un quadro di precarietà che andrebbe immediatamente superato e che sicuramente vedrà il nuovo vertice della SOGIN impegnato ad adottare tutte le misure necessarie a gestire le attività di messa in sicurezza e di custodia dei siti e dei materiali in essi presenti in termini di maggiore accortezza, tanto da offrire le ordinarie e minimali garanzie richieste dalle norme internazionali in materia.

il sottosegretario Bubbico per le risposte e manifesto anche una relativa soddisfazione perché, al di là della

nelle considerazioni finali, mi pare vi sia, con riferimento alle prime misure contenute nella finanziaria e

nelle interrogazioni. Si tratta della conferma, cioè, di una gestione gravemente deficitaria, sotto tutti i punti di vista, di una società come la SOGIN in un rapporto con un'altra società di estrema importanza strategica come l'ENEA. Noi constatiamo, anche attraverso

impianti, che gli interventi risolutivi sono oggetto di decisioni recenti e perfino successive alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione. Ci rendiamo conto che noi, come Paese, e i lavoratori interessati siamo stati esposti a rischi gravissimi. Quando il Sottosegretario parla di ripristino di condizioni ordinarie e minimali vuol dire che eravamo in una condizione di estrema pericolosità. Quello che è peggio, sottosegretario Bubbico, è che i lavoratori e i rappresentanti sindacali che hanno segnalato, sia in occasione di incontri sindacali con la direzione aziendale,

nel senso del disconoscimento dei loro valori professionali. Tra l'altro, erano stati già, nei cinque-sei anni precedenti, discriminati a favore e a vantaggio

impianti e situazioni come quelle che si sono determinate. Peraltro, siamo in presenza di personale non qualificato, non preparato, senza il

diretti, sia mettendo da parte i responsabili dei progetti e coloro i quali avevano la titolarità e le qualificazioni professionali adeguate,

come mai la SOGIN avesse affidato a trattativa privata alla società ELECTRON, ancorché del gruppo Finmeccanica, lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento del quadro elettrico.

sempre di competenza dell'ENEA e della Casaccia, non ha alcuna competenza in materia di quadri elettrici.

di un difetto di realizzazione dei collegamenti nel quadro elettrico. È andata bene così, ma se per caso la porta blindata fosse stata chiusa dall'operatore che doveva realizzare l'intervento, non soltanto costui sarebbe stato disintegrato, ma l'intera costruzione sarebbe esplosa in ragione della massa di 36 bombole di anidride carbonica e dell'attivazione di processi che vedono interessato direttamente il plutonio nel sito specifico della Casaccia. A me fa piacere che il Governo abbia affidato alla SOGIN anche la revisione di compiti e di procedure e mi auguro che questo possa portare rapidamente a una messa in sicurezza degli impianti, all'intervento relativo alle centrali nucleari in dismissione, che rappresentano un altro degli elementi di possibile contaminazione.

sono riuscito ad avere un collegamento, nel quale, tra l'altro, mi è stato detto che si trattava di un banale incidente, che era esplosa una bombola, ma che tutto andava bene. Contemporaneamente, invece, mi arrivavano le informazioni dei lavoratori, dei tecnici dell'impianto che mi raccontavano come stavano realmente le cose, comprese le verifiche che i Carabinieri e i Vigili del fuoco, appena arrivati, avevano iniziato a fare non soltanto sull'impianto, con

secrezioni mucose dei lavoratori. Prendo atto, con soddisfazione, della completezza dell'informazione e auspico che sugli sugli elementi segnalati vi possa essere, anche in Commissione, un'informazione più completa che riguardi non solo lo stato di revisione dei compiti, ma anche la verifica dell'opportunità che la SOGIN, in quanto tale, continui a essere referente prioritaria dell'ENEA o non si debba, nel quadro della sua riorganizzazione, puntare ad un altro assetto.

e al prelievo venatorio», la seduta antimeridiana di martedì 20 febbraio, per la quale il calendario prevedeva, appunto, il seguito della discussione generale medesima,